apre una nuova finestra"). Colleghi, è arrivata la seguente richiesta di cui do lettura, che è preliminare al prosieguo dei nostri lavori: «I sottoscritti senatori, ai sensi delle disposizioni regolamentari di cui al comma 4 dell'articolo 56, considerato che le Commissioni finanze e lavoro riunite in data 22 luglio hanno concluso l'esame del disegno di legge atto Senato n. 890, di conversione in legge del decreto-legge n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, considerato che nel cronoprogramma della riunione dei Capigruppo del 16 luglio era stata fissata come data ultima per l'approvazione del presente disegno di legge di conversione, vista l'effettiva necessità ed urgenza di interventi finalizzati a promuovere misure di contrasto alla crescita esponenziale del fenomeno della disoccupazione dovuta alla grave congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese, chiedono di procedere immediatamente alla discussione e votazione dell'Atto Senato n. 890». La richiesta è sottoscritta dal senatore Bitonci e da altri senatori. Si tratta sostanzialmente

essendo esaurita la discussione generale del provvedimento affrontato questa mattina, l'atto Senato n. 896 ed essendo stati acquisiti tutti i prescritti pareri, non vede la necessità di tale inversione. Tuttavia, trattandosi di una importante motivazione della richiesta, ritengo si possa procedere ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, quindi con l'intervento di un oratore a favore e uno contro, per poi rimettere all'Assemblea

C'è un preciso riferimento al comma 4 e non al comma 3 dell'articolo 56. Diversamente, non ci sarebbe stata neanche la necessità Mi scusi, presidente Calderoli, ma il comma 4 fa riferimento

Ci sono due argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna: l'Atto Senato n. 896 e l'atto Senato n. di cui è stata chiesta l'anticipazione. Non è previsto l'inserimento di un nuovo argomento all'ordine del giorno, ma solo l'inversione, che è oggetto della richiesta che ho testé letto, se non ho capito male.

Ma è già all'ordine del giorno. Non abbiamo iniziato la discussione; la discussione è stata sospesa nella seduta di stamattina, che si è conclusa. Oggi abbiamo un nuovo ordine del giorno, che reca due punti: punti: il seguito della discussione del disegno di legge n. 896 e l'esame del disegno di legge n. 890, che è già inserito all'ordine del giorno. Per cui la inviterei, se ritiene, ad intervenire, a termini di Regolamento, a sostegno della richiesta.

al tema del lavoro. Tutti quanti in questo momento vedono e vivono delle difficoltà nei loro territori: aziende che chiudono, lavoratori che non hanno contratti o contratti a tempo determinato, quindi con difficoltà di avere prospettive future, aziende che non hanno finanziamenti o supporti per poter dare risposte. Noi siamo convinti che il disegno di legge n. 890 debba essere discusso con priorità assoluta, per dare risposte al Paese, per non accettare assolutamente un aumento di un punto dell'IVA,

migliaia di giovani, di famiglie e di imprenditori che aspettano risposte e hanno diritto di averle da questo Governo. Noi vogliamo quindi che ci siano risposte in base a una finanziaria concreta, corretta e responsabile. Dobbiamo dare risposte ai cassintegrati e agli esodati

Si parla di IVA su qualche cosa che i nostri produttori non riusciranno a vendere. Si parla di anticipazioni di IRPEF, di IRES e di IRAP per delle aziende che non produrranno più niente, se non date delle risposte concrete. Quindi noi vogliamo che i giovani abbiano lavoro

nessuno ovviamente intende sminuire il valore dell'urgenza richiamata adesso dalla senatrice Bellot, ma faccio osservare alcune cose. Questo provvedimento è in calendario dalla scorsa settimana, secondo un calendario approvato da tutti i Gruppi parlamentari, e le urgenze richiamate adesso dalla collega Bellot non sono urgenze di oggi, ma sono purtroppo urgenze di mesi. Entrambi i provvedimenti sono conversioni in legge di decreti, quindi le misure che contengono sono già a tutti gli effetti legge. Le modifiche che il Parlamento potrà apportare in sede di conversione sono certamente importanti, ma non incidono né sullo slittamento dell'IVA, previsto dal decreto-legge

nel momento dell'incardinamento di questo provvedimento nella giornata di ieri, nella quale i colleghi non hanno ritenuto di chiedere un'inversione o una diversa definizione del calendario dei lavori. Ci sembra che la priorità sia di concludere rapidamente l'esame del provvedimento in titolo, la cui conversione comunque darà solidità alle risposte a un'altra emergenza, quella delle carceri che scoppiano e che mettono l'Italia in una condizione di violazione di tutte le normative internazionali (ricordo che abbiamo già subito una condanna da parte della Corte di giustizia europea). Si tratta, quindi, di procedere senza indugio alla votazione degli emendamenti e alla conversione del decreto-legge, e immediatamente dopo provvederemo provvederemo a discutere e a convertire il decreto in materia di lavoro e di IVA, che è stato licenziato ieri sera dalle Commissioni competenti. Pertanto, siamo contrari alla proposta di inversione

1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, - preso atto delle assicurazioni del Governo circa il modesto impatto sulle strutture pubbliche di assistenza e cura del maggior ricorso agli arresti domiciliari, e in ogni caso circa la capacità di tali strutture di far fronte a maggiori impegni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; - preso atto altresì della capienza attuale della contabilità speciale di cui al capitolo n. della quale si vale il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché della pianta organica del medesimo ufficio; esprime, per quanto di propria competeva, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sostituire le parole «sul capitolo 5421 assegnato alla» con le seguenti: «sulla»; all'articolo 4, comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.1, 4.9, 4.9/3, 4.9/3 (testo 2), 4.0.1, 5.1, 5.1, 5.1/1 e 5.200. Sull'emendamento 4.3, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo la parola «assume», delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,". Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti».

Signora Presidente, intervengo con riferimento al parere che è stato espresso dalla Commissione bilancio. Devo dire la verità: non comprendo la ragione

l'emendamento 4.9 non implica alcun impegno di spesa e prevede semplicemente la procedura e la regolamentazione per l'eventuale permuta di beni immobili nella disponibilità del Ministero della giustizia, sì da poter realizzare ulteriori immobili o riammodernare gli immobili già esistenti.

delle modifiche di natura letterale, cioè si tratta sostanzialmente di un'operazione, se vogliamo, di *drafting* allargato, con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge, nei cui confronti c'è piena adesione da parte della Commissione bilancio. non riesco a comprendere la ragione per la quale, stante la sintonia con l'articolo 81 della Costituzione dell'articolo 4 del decreto-legge, debba ritenersi in violazione dell'articolo 81 della Costituzione un emendamento che recita quanto segue: «(...) sostituire le parole: "realizzati all'esito delle procedure di cui ai precedenti commi" con le seguenti: "di cui alle procedure del presente articolo"». Non vi è chi non veda come questa sostituzione non ha alcuna nessuna incidenza sotto il profilo della copertura finanziaria e che, se del caso, un'illegittimità ai fini dell'articolo 81 della Costituzione può esistere solo se esiste analoga illegittimità dell'articolo che si va ad emendare con l'emendamento 4.9/3. Ed è inutile, signora Presidente, che io continui a leggere il testo degli emendamenti a cui facevo riferimento. Ora, non vi è dubbio che questi articoli verranno trattati successivamente, per cui ritengo che possiamo tranquillamente andare avanti, ma sarebbe sommamente opportuno che dalla Commissione bilancio arrivasse una chiarificazione che non si sostanzi, come accade, nel mero richiamo all'articolo 81 della Costituzione, perché così com'è davvero non è molto comprensibile. Senatore Palma, come lei ha osservato, si tratta di pareri che si riferiscono ad emendamenti che affronteremo successivamente. In ogni caso, è preliminare procedere alla valutazione della richiesta

Ai cittadini dobbiamo dare risposte congruenti anche rispetto all'aspettativa di sicurezza, in un momento in cui tutto diventa più difficile; una difficoltà che non nasce solamente dalla crisi economica, ma anche da una crisi di identità, una crisi di identità, che sta colpendo tutto il Paese. Ne abbiamo potuto parlare prima, in sede di 14a Commissione, quando ci siamo trovati a confrontarci con i nostri colleghi eurodeputati. In quella circostanza abbiamo appreso - come peraltro già sapevamo - come le politiche della stessa Unione europea siano molto differenti da Paese a Paese.

che consenta a noi di aver chiaro che quello che stiamo facendo o andremo a fare possa avere un significato non solo estemporaneo, ma anche compiuto, che garantisca ai cittadini maggiore sicurezza e maggiore certezza. Questo avviene in Italia oggi, ma avviene anche in altri Paesi europei. Non possiamo trascurare il fatto che, in questa circostanza, non possiamo operare in maniera disgiunta rispetto

senza creare insicurezza nel nostro tessuto sociale. Altri Paesi europei hanno già affrontato questo problema? Non lo so: probabilmente sì, probabilmente altri lo stanno facendo con altre modalità. Noi dobbiamo certamente approfondire questo tema; la discussione degli articoli oggi potrebbe, invece, tranciare ogni possibilità di approfondimento, un approfondimento che non può essere negato a una sede parlamentare, nella quale qualsiasi qualsiasi voce rappresenta quella di tanti altri cittadini. Credo di rappresentare, ad ogni buon diritto, la voce di chi vuole sicurezza e non chiede in questo momento una discussione finalizzata semplicemente a soddisfare un'esigenza del Governo: quella di approvare un decreto-legge

Il mio consenso andrà nella direzione della proposta del senatore Santangelo.

anche chi è contrario a questo provvedimento deve condividere con l'Aula la responsabilità di fare in modo che gli effetti del decreto-legge, che già sono in corso, siano valutati attentamente. Noi li valutiamo positivamente, ma anche chi li valuta negativamente ha la responsabilità di condividere con noi un *iter* che consenta al Governo di veder convertito

dalla depenalizzazione di alcuni reati minori, dal costruire nuove carceri (cosa che si sarebbe potuta fare negli anni passati e avrebbe dato magari stimolo all'economia e alle imprese a livello locale), dalla ristrutturazione di quelle esistenti: operazioni che sono state sempre rinviate, non si sa per quale motivo. Forse, anzi, un motivo c'è: ogni volta che c'è un'emergenza è possibile derogare alle regole ordinarie;

non possiamo misurare i reati da punire in funzione degli spazi che abbiamo per ma dobbiamo misurare gli spazi affinché ci sia una detenzione dignitosa per tutti coloro che devono essere puniti per aver commesso un reato. Pertanto, piuttosto che dell'esecuzione della pena andrebbe effettuata una revisione sostanziale di alcuni reati

recuperare un minimo di coerenza rispetto alle cose che diciamo e che facciamo. Prima ci viene detto che c'è la necessità di inserire all'ordine del giorno un provvedimento urgente, cioè quello sul lavoro. lavoro. Adesso i colleghi della Lega introducono un elemento di dilazione della discussione per cui quel provvedimento che era così urgente un quarto d'ora fa non lo è più. Penso sia

penso però che, al di là delle motivazioni che sono state addotte dal rappresentante della Lega e poi dal senatore Crimi, la proposta così come formulata dal senatore

sulla base di un ragionamento logico, la possibilità di valutare se la richiesta può essere da noi votata favorevolmente o meno.

però si richiama una norma del nostro Regolamento in virtù della quale si formula una determinata richiesta. Ribadisco, pertanto, l'esigenza di conoscere effettivamente quale motivazione si accompagna ad una richiesta che, peraltro, in questo caso brucerebbe il provvedimento perché, come sappiamo, trattandosi di un decreto‑legge non ci sarebbero più i tempi necessari per

molto più palesemente discordanti da quelli che segnala la nostra Carta costituzionale. Nel caso specifico, peraltro, parliamo di condizioni

che, pur condividendo io in linea di principio l'idea secondo la quale è naturalmente più giusto dare centralità al Parlamento e quindi evitare la decretazione d'urgenza ed intervenire attraverso la classica procedura parlamentare dell'Aula, nel caso specifico vorrei che non si dimenticasse una sentenza della Corte europea di Strasburgo, la cosiddetta sentenza pilota Torreggiani. Questa sentenza obbliga il nostro Paese ad intervenire sul tema del sovraffollamento nelle carceri e considera inumano e degradante il trattamento a cui il nostro Paese sottopone i suoi detenuti all'interno delle patrie galere. Pertanto, vorrei che quest'Aula, sempre molto attenta a quanto arriva dal Nord Europa, anche su questo argomento fosse sensibile.

a valutare le opportune iniziative tese a far sì che una qualsiasi delle autorità competenti: *a)* non disponga e non consenta

che permetta la tortura in carcere deve essere punita come qualsiasi altro cittadino, altrimenti fa sorridere la scritta «La legge è uguale per tutti». Invito quindi il Sottosegretario a

la contrarietà sull'ordine del giorno G100 era collegata alla responsabilità oggettiva in capo ai vertici delle amministrazioni giudiziarie e penitenziarie prevista dall'ordine del giorno nella originaria formulazione. Così come riformulato, l'ordine del giorno corrisponde pienamente agli obiettivi del decreto-legge oggi all'esame del Senato e quindi non possiamo che esprimere parere

Si tratta di un tema delicato, affrontato più volte in quest'Aula del Senato, e anche alla Camera, riguardante i servizi sanitari a tutela delle persone detenute: l'assistenza specialistica ambulatoriale, la valutazione dello stato di malattia e anche di morte dei detenuti, l'assistenza continuativa per le persone affette da patologie croniche e la questione degli ospedali psichiatrici giudiziari. Non mi sembra che ci sia nulla di sconvolgente. Se la collega Granaiola non ritiene di dover accettare l'accoglimento dell'ordine

Signora Presidente, visto che il Governo non è ostile a questo ordine del giorno, vorremmo chiedere se, riformulandolo, c'è la possibilità di addivenire ad un parere favorevole.

Grazie,

intervengo brevemente. Il nostro primo emendamento, l'1.1, è volto alla soppressione dell'intero articolo 1, per le motivazioni già esposte in discussione generale dai colleghi, visto che riteniamo queste norme assolutamente contrarie e destabilizzanti per il nostro sistema.

che all'articolo 10, lettera *e)*, stabilisce che, tutte le volte in cui la norma si aggiunga al comma 1, assuma la numerazione 01. Al contrario, nel testo da noi utilizzato non c'era la numerazione dei commi, quindi avevamo ritenuto comma 1 quello che di questo difetto di coordinamento tra un testo legislativo che recava la numerazione dei codici e un altro che invece non la recava,

il parere è favorevole

caso invitiamo al ritiro ed eventualmente ad elaborare un ordine del giorno su questo punto, poiché la materia è già regolamentata

Per quanto riguarda l'emendamento 1.52 della Commissione, il parere è favorevole, a condizione che venga così riformulato:

"423-*bis*, 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis* del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti

il relatore ha spiegato le ragioni per le quali ha espresso un parere contrario all'emendamento 1.38 della Commissione. Vi è sostanzialmente un invito al ritiro. L'emendamento deve, quindi, intendersi ritirato.

Signora Presidente, chiederei un attimo di attenzione perché la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento approvato dalla Commissione

andremmo a dire che si sospende l'esecuzione per un condannato per furto che abbia la doppia aggravante o più di due aggravanti. se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, questa è un'aggravante. Se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito,

è stata discussa proprio durante la passata legislatura; essa riguardava le povere persone anziane che, davanti agli istituti di credito, vengono derubate della pensione o di quello che vanno a prelevare. Credo che sarebbe un errore gravissimo togliere questa possibilità della sospensione; peraltro ci sono due o più aggravanti.

Grazie,

Grazie,

di sorveglianza una misura che da una parte consenta l'allentamento della pressione detentiva ma, dall'altra, mantenga un controllo, seppure a distanza, sul detenuto. Mi si dice

circa la concessione del beneficio. Credo sia una norma di buonsenso, un incentivo ad utilizzare strumenti di controllo elettronico, che sono

giustizia*. Confermo il parere contrario sull'emendamento, che attesta il fatto che trattasi di materia già regolamentata dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario e dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

Castello nella fila in alto alla mia sinistra, si accendevano tutte e cinque le luci, mentre sono presenti quattro senatori. Probabilmente vi è un problema nel tabellone. *(Applausi

sul piano strettamente formale faccio presente al senatore Caliendo che il testo dell'emendamento è stato portato in Aula dalla Commissione, conseguentemente fuoriesce dalla disponibilità di chi lo aveva presentato nella fase emendativa, durante i lavori della Commissione.

ovvero di decidere sull'istanza relativa alle misure alternative di cui agli articoli 47 e via dicendo, ivi compresa la detenzione domiciliare. Con riguardo alla norma cui si correla l'emendamento 1.52, si dice che questo ordine di esecuzione non può essere sospeso in determinati casi,

nel testo originale proposto dalla Commissione erano inseriti anche, come reati per cui è vietata la sospensione dell'ordine di esecuzione, i delitti di furto pluriaggravati; nella riformulazione del Governo, invece, vengono inseriti solo i reati di furto di cui all'articolo 624-*bis*, cioè il furto in appartamento ed il furto con strappo, le due tipologie di furto sicuramente più gravi rispetto alle altre tipologie previste dagli articoli 624 e 625.

dal senatore Caliendo personalmente non mi convince. Non possiamo infatti che avere riferimento alla oggettiva gravità dei reati, e quando il senatore Caliendo pensa all'indubbio aumento della criminalità che deriva dalle situazioni di crisi economica - questa è una costante dei ragionamenti di economia - immagino che probabilmente faccia riferimento non a quei reati di particolare efferatezza, ma a reati correlati alle effettive necessità dei cittadini derivanti, per l'appunto, dalla crisi economica.

non ho bisogno di una sospensione. Se ho capito bene, non avendo il testo della riformulazione, viene solo espunto

Grazie, di minacce gravi. A tutti noi capita, per la nostra attività politica, di ricevere minacce. A molti di noi è capitato, ma considero questo documento gravissimo per le minacce che contiene e per la firma, con una stella a cinque punte. È una cosa molto grave. Desidero, a nome di tutti i senatori del Partito Democratico, esprimere grande solidarietà

ci facciamo garanti affinché ciascuno di noi possa dire quello che pensa, sempre, in ogni circostanza, e tutti noi siamo al fianco di chiunque di noi dovesse dire qualcosa che anche non condividiamo. La libertà del Parlamento è infatti la cosa più sacra, il marchio più sacro di una democrazia, e tutti noi, insieme, ci impegniamo per tutelarla. *(Applausi anch'io voglio associarmi alle parole del senatore Zanda. Vorrei solo dire che finora la battaglia che Stefano Esposito ha condotto, qualche volta anche da solo, in Piemonte, in Provincia di Torino, in Val di Susa, non è conosciuta da tutti. Vorrei ricordare che questi episodi non avvengono a caso ma: sono il frutto di intimidazioni e tentativi di conculcare la libertà di pensiero e di azione di una persona che da anni si sta battendo per un'opera pubblica di vitale importanza per Torino, il Piemonte e l'Italia non sempre è stato adeguatamente supportato da tutti noi, che - pure - nelle Aule istituzionali questo provvedimento lo abbiamo votato e sostenuto. quindi che tutti comprendano veramente, fino in fondo, qual è il clima in cui chi è favorevole a quell'opera si trova a dover vivere, per poterla sostenere e spiegare all'opinione pubblica e alle popolazioni. Questo riguarda sia chi è in prima fila come politico a sostegno dell'opera, sia chi in quei luoghi si è opposto in maniera davvero forte alle intimidazioni ed alle violenze che sono state perpetrate nei confronti di uomini delle forze dell'ordine, dei sindaci favorevoli, degli imprenditori e dei cittadini che l'hanno sostenuta.

settimana. Ormai gli osservatori non capiscono più le ragioni di una protesta che sta diventando qualcosa di diverso e di violento.

sia importante discutere tra le parti, ma la discussione deve sempre essere civile e non portata avanti, come sta avvenendo in questi giorni, in maniera violenta e cruenta.

armi, bastoni e maschere antigas, come se partecipassero ad un vero e proprio assalto, e alle forze dell'ordine che difendono i nostri diritti in quella zona. Grazie, Stefano, per il tuo lavoro.

Detto questo, fatta salva questa critica politica, esprimo la totale solidarietà del mio Gruppo al senatore Esposito, in quanto nessuna dichiarazione politica di un parlamentare della Repubblica,

vedere. La solidarietà di Sinistra Ecologia e Libertà al senatore Esposito è ovviamente incondizionata.

presente con estrema franchezza che in Val di Susa ormai l'opposizione alla realizzazione dell'infrastruttura di cui stiamo parlando non è solo un esercizio di democrazia, anzi devo dire che non è più un esercizio di democrazia. Le manifestazioni, sia sul territorio che nei confronti di coloro che hanno espresso e si esprimono favorevolmente all'opera, assumono una connotazione forte di grande intimidazione, di minaccia all'integrità fisica delle persone: si tratta di situazioni eversive, e chi ha la mia età sa quanto siano simili a quelle già viste in altre epoche nel nostro Paese. Quindi, la solidarietà delle parole è importante, ma è necessario mettere in atto ogni iniziativa volta a rimuovere questo atteggiamento ribellistico, che comporta un grandissimo disagio economico per le popolazioni di quei territori, che ritarda la realizzazione di un'opera importante per il nostro Paese, che costa in termini economici e finanziari alle istituzioni pubbliche che sono chiamate al mantenimento dell'ordine su quel territorio. Da questo accorato impegno di solidarietà al collega deve venire anche una manifestazione concreta di potenziamento della presenza dello Stato nel territorio,

è ammesso qualsiasi tipo di ricorso. Riteniamo invece che in una democrazia ognuno debba poter esprimere il proprio pensiero, le proprie opinioni e le proprie

comunque la piena solidarietà del nostro Gruppo al collega Stefano

erano le Brigate Rosse, al cui simbolo si è fatto riferimento. Ci corre però l'obbligo di porre l'attenzione su gravissimi e violenti fatti svoltisi in Val di Susa il 19 luglio, che riguardano un'attivista di 33 anni, Marta Camposana, del movimento No

Esposito. Credo sia responsabilità di tutte le forze politiche evitare che l'aggressività o la violenza verbale, che sono così diffuse, si trasformino gradualmente in qualcosa di molto più serio e preoccupante.

Il testo dell'emendamento 1.52 della Commissione recitava così: «*Al comma 1, lettera* b)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

Qual è la conseguenza? Che la lettera *b)* e la lettera *c)* sarebbero rimaste in vita, rispetto al testo del decreto‑legge che invece le sopprimeva. Il Governo presenta una riformulazione diversa

La differenza è molto semplice. semplice. Con il testo della Commissione, sarebbero rimaste in vita le lettere

nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare» - ed è logico che sia così, perché già sono in stato di custodia cautelare - nei confronti dei condannati ai quali si stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale», cioè i recidivi specifici infraquinquennali. Con il testo del Governo, invece, si ritorna al passato del decreto‑legge e sostanzialmente muoiono definitivamente le lettere *b)* del comma 9, contrariamente a quello che era stato approvato in Commissione e che era oggetto dell'emendamento del senatore Caliendo.

contrariamente a quello che era stato deciso in Commissione, la sospensione può essere disposta nei confronti dei recidivi specifici infraquinquennali. Secondo il testo della Commissione e dell'emendamento riformulato - che noi immaginavamo fosse riformulato in quel senso - tutto questo non è possibile. Pertanto, arrivando alla conclusione, gradirei capire dal Governo

dimostra che va affrontata in maniera adeguata. Non credo che la sede più adeguata per affrontare questo tema sia l'Aula del Senato. Tra l'altro, ricordo che già in Commissione c'è stato un

e alla possibilità di concedere o meno determinati benefici, credo che proprio per trovare il punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza sociale e le esigenze segnalate nella normativa che stiamo per approvare, sia opportuno un approfondimento tra i vari Gruppi che compongono il Senato e il Governo, proprio per evitare nella maniera più assoluta qualsiasi contrasto e soprattutto incomprensioni all'esterno dell'Aula. Chiedo, quindi, un accantonamento. [**Presidenza sono d'accordo con il senatore Casson; credo sia bene fare una piccola verifica, con calma, perché su questo punto ci sono esigenze diverse da compenetrare e da rendere compatibili. Credo non sia bene procedere in ordine sparso.

Signor Presidente, la domanda che ha rivolto il senatore Palma al Governo credo sia di assoluta rilevanza e piacerebbe a tutta l'Assemblea, e non solo agli addetti ai lavori,

Nel momento in cui chiede di parlare, il Governo deve essere messo in grado di esprimersi, e quello che ha chiesto il senatore Palma mi sembra assolutamente rilevante.

se si accantona questa materia va accantonato anche l'ordine del giorno G1.100.

50-*bis* concerne la semilibertà, che può essere sempre concessa a coloro che sono recidivi specifici reiterati, ma ovviamente, rispetto a chi è condannato per la prima volta, è specificata una serie di condizioni.

Credo che andare a ritoccare queste norme significhi abbassare il livello di deterrenza per chi delinque.

Una volta richiamata la lettera *a)* e fatto il riferimento alla quota edittale di quattro anni di reclusione, la stessa modificazione doveva riflettersi sulla lettera *b)*. Per cui la lettera *b)* viene modificata nel modo seguente: «nei «nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena».

alla materia dei permessi premio e della semilibertà, non vi siano limitazioni concernenti le quote di pena che devono essere espiate, per i recidivi aggravati e reiterati, differenziate rispetto alle quote di pena richieste per i cosiddetti delinquenti primari: costoro, trascorsa la metà della pena, infatti, potrebbero godere dei benefici in questione, ossia

(recidivi aggravati e reiterati), il beneficio possa essere concesso soltanto una volta. Cadrebbe, quindi, il divieto di concessione soltanto per una volta del beneficio per questa categoria di delinquenti. In Commissione vi è stato contrasto: per questa ragione non esprimo un parere e mi rimetto all'Assemblea. Mi permetto, però, di notare una sola circostanza, tra le tante che potrebbero essere richiamate: la materia dei permessi premio e della semilibertà non incide sull'eccesso di popolazione detenuta. I soggetti ammessi all'uno ovvero all'altro beneficio continuano, comunque, sia pure con modalità differenziate, ad essere soggetti detenuti. Sostanzialmente, quindi, nel mitigare le disposizioni limitative per i recidivi di cui al quarto comma dell'articolo 99,

«I detenuti e gli internati di norma possono essere» con le seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai detenuti e agli internati». Richiamiamo cioè espressamente tutta la disciplina del lavoro all'esterno con riferimento a questo tipo

al numero 4) della lettera *b)* il comma 9 è sostituito dal seguente: «La condanna per il delitto di cui al comma 8 importa la revoca del beneficio». Si tratta sostanzialmente della condanna per il delitto di evasione.

hanno creato oggettivamente un po' di confusione tra Commissione e Governo in ragione del fatto si faceva riferimento a due testi diversi.

le circostanze, forse la soluzione migliore sarebbe di rinviare a domani il seguito della discussione e delle votazioni, così da consentire al Governo e alla Commissione di realizzare i dovuti approfondimenti in ordine alle varie riformulazioni.

Presidente, volevo stigmatizzare un fatto accaduto in questi giorni e che riguarda la mia Regione di provenienza, la Basilicata. È troppo recente il ricordo dell'uso strumentale, e direi anche molto disinvolto, della funzione giurisdizionale. Mi viene subito alla mente l'esperienza vissuta in queste recenti consultazioni politiche con il dottor Ingroia. Non so se voi ricordate la questione delle toghe lucane, quel megaprocesso che ha fatto un po' la storia e la cronaca del nostro Paese, dove non bagatelle ma reati seri, come corruzione e associazione a delinquere, vedevano sul banco degli imputati i magistrati del palazzo di giustizia di Potenza e di Matera, 30 indagati. Quel processo non è neanche iniziato, perché l'impianto accusatorio del pm De Magistris non riuscì neppure ad arrivare in dibattimento. "Archiviazione", sentenziò il gip, e trenta persone si ritrovarono dall'oggi al domani con una reputazione che gli organi di stampa erano riusciti ad infangare in modo indelebile; e tutto questo dovuto

cui si era individuato per la prima volta, con una certa serietà imprenditoriale, in una realtà come quella meridionale, un insediamento di porto turistico che aveva messo in cantiere un'attività estremamente importante, soprattutto in un momento delicato quale quello che viviamo: anche il processo di appello di Catanzaro si è concluso con di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Questo processo ha un risvolto ancora più importante dal punto di vista economico, perché non posso non denunciare che,

alla possibilità di arricchimento del territorio. La domanda che mi pongo - e che volevo rivolgere anche ai capigruppo

ci ha fatto praticamente capire che attraverso questi falsi processi si possono costruire delle carriere politiche, volevo chiedere ai Capigruppo se non sia il caso

di questa occasione per stigmatizzare un evento che ancora una volta lascia molto stupefatti, per così dire. Ho avuto più volte occasione di come spesso la filosofia dei tagli lineari faccia veramente dei disastri molto più gravi di quei problemi che vorrebbe risolvere. Faccio riferimento al tribunale di Modica, della cui chiusura ho cercato di coinvolgere molti dei nostri senatori, che insieme a me sono venuti nella città di Modica per vedere cosa si sta compiendo con quest'atto diretto a chiudere un tribunale che è stato inaugurato pochi anni fa e che è costato soltanto 12 milioni di euro. Tutto questo per risparmiare e concentrare l'attività giudiziaria nel vicino capoluogo, la città di Ragusa. Ebbene, adesso (ed è per questo che intervengo, perché io ho sollecitato la Commissione giustizia, ho presentato interrogazioni, i colleghi sono venuti a Modica e si sono resi conto della

chiediamo altri fondi al Ministero per andare a rinforzare delle strutture che naturalmente non possono essere adeguate per accogliere tutto il lavoro che riguarda entrambi i tribunali.

Signor Presidente, abbiamo già in qualche modo indirettamente toccato, esprimendo la nostra solidarietà al collega Stefano Esposito (solidarietà alla quale naturalmente mi associo), un tema che mi mi proponevo di riportare all'attenzione dell'Aula. Mi riferisco agli episodi che abbiamo dovuto ancora in questi giorni registrare in Val di Susa, episodi che, purtroppo, non è la prima volta che ci tocca ricordare in quest'Aula, e temo non sarà neppure l'ultima. Nel commentare quello che ormai reiteratamente accade in quella valle, nel raccontare degli episodi di aggressione e violenza organizzata e sistematica di cui sono fatti oggetto gli operai dei cantieri, i tecnici del cantiere e le forze dell'ordine che sono a presidiare il regolare svolgimento delle operazioni, ogni volta ci siamo trovati a dire dire che si è davanti a un pericoloso salto di qualità, rispetto al quale è importante produrre da parte delle istituzioni un corrispondente salto di qualità sul fronte

le frange violente che pure si annidano in valle nel movimento No TAV ormai per consuetudine appaltano a gruppi provenienti dall'esterno il compito di scatenare le azioni di carattere insurrezionale e di guerriglia. Il paradosso è che in quella valle si sta registrando un fenomeno per cui un senatore della Repubblica, un rappresentante delle istituzioni che voglia andare in quelle zone a sostenere in un libero libero confronto democratico le ragioni per realizzare l'opera non lo può fare, mentre coloro che si rendono protagonisti, arrivando da ogni parte d'Italia e d'Europa, delle scorribande che conosciamo possono agire liberamente. Credo Credo che lì sia ormai evidente che c'è una questione su tutte che si è aperta: la questione di ripristino della legalità democratica. Prima ancora

l'agibilità democratica. Arriverà alla Presidenza del Senato, come alla Presidenza della Camera, la richiesta di un gruppo di sindaci della valle che chiedono che le le forze parlamentari si ritrovino lì per celebrare una giornata sul tema della convivenza democratica, non sul tema dell'opera, per dare il segnale... *(Il microfono Signor Presidente, colleghi senatori, mi riallaccio a quanto già detto prima, e quindi, come Movimento 5 Stelle, condanniamo qualsiasi tipo di attacco o minaccia, ma chiedo altrettanta solidarietà in riferimento a quanto accaduto alla signora Marta Camposana. Mi riferisco ai gravissimi e violenti fatti svoltisi in Val di Susa il 19 luglio scorso e che riguardano un'attivista di 33 anni, appunto Marta Camposana, del movimento No La donna ha dichiarato: «Da quando mi hanno fermata a quando mi hanno portato all'interno del cantiere sono stati dieci minuti di follia. Ho ricevuto una manganellata in faccia, mi hanno toccato nelle parti intime e mi hanno insultata». Ovviamente tale ricostruzione dei fatti necessita un approfondimento in sede giudiziaria, che auspichiamo. Ma ora siamo qui a ricostruire quello che è avvenuto dopo. Ebbene, leggiamo sbigottiti il *tweet* e le successive dichiarazioni di tono similare di un rappresentante delle istituzioni, il senatore Stefano Esposito, poi ripresi dai giornali, che afferma riferendosi alla donna: «Parte da Pisa per andare a fare la guerra allo Stato, prende giustamente qualche manganellata e si inventa di essere stata molestata #bugia». Il senatore Esposito, senza la benché minima traccia di pudore o vergogna, dichiara apertamente non solo di ritenere giuste le manganellate che la donna riferisce di aver subito, ma si pronuncia come un giudice senza averne il titolo, dichiarando addirittura che la donna mente, inscenando una molestia inesistente. Questo ci porta alla memoria tutte quelle volte che le donne hanno subito violenza e non hanno ricevuto giustizia, perché degli uomini troppo vili per ammettere la loro stessa viltà addossavano alle donne ogni colpa, negando l'evidenza dei fatti. Come donne e cittadine ci sentiamo indignate e ci chiediamo come sia possibile giustificare e legittimare ogni forma di violenza e maltrattamento. Le parole di Esposito, di sostegno all'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine proprio contro una donna, risultano ancora più assurde e contraddittorie da parte di chi ieri sosteneva con il proprio voto sosteneva con il proprio voto la Convenzione di Istanbul. Il senatore Esposito rappresenta, con le sue parole, la concretizzazione dinanzi ai nostri occhi e a quelli dei cittadini della manifestazione più insidiosa della violenza, intesa come fenomeno culturale, poiché in modo malcelato il messaggio che ci viene offerto è terribile nella sua viltà. Secondo Esposito, quindi, in presenza di un'opinione di dissonanza è legittima una reazione violenta, ancor più se l'opinione proviene da una donna. Allora la risposta deve essere muscolare e maschilista. A questo punto, riteniamo necessario capire se questo pensiero di istigazione alla violenza nei confronti di chi dissente, soprattutto nei confronti delle donne, è un pensiero individuale del senatore Esposito o se è condiviso

Grazie, presidente l'intervento che intendo fare vuole portare all'attenzione dell'Aula del Senato alcuni episodi che sono accaduti in questi giorni e che ritengo debbano essere oggetto di riflessione da parte di tutti, soprattutto da parte del legislatore. Sembra un intervento in controtendenza con quanto stiamo discutendo in queste ore, ovvero la depenalizzazione. Però ha destato parecchio sconcerto nelle rispettive comunità locali quanto accaduto a Gorgonzola e quanto accaduto a Brebbia, dove, in due circostanze differenti ma assolutamente simili, due giovani sono stati travolti da pirati della strada e, in ciascuno dei due casi, abbandonati senza soccorso (omissione di soccorso). Ho partecipato l'altro giorno, insieme a tante persone, insieme al sindaco del paese e insieme a tanti cittadini, alla manifestazione che si è tenuta a Brebbia, in provincia di Varese, per dire in maniera silenziosa alla famiglia del piccolo Alberto che tutta la comunità si stringeva vicina in questa circostanza veramente difficile. È stata una manifestazione molto civile e molto intensa e commovente, nella quale non c'è stata alcuna espressione di odio. C'è stata invece una grande stretta attorno alla famiglia, per far sentire la solidarietà di una comunità. Ma da persona a persona raccoglievo un'istanza, che desidero portare all'attenzione e ritengo importante che sia tenuta in conto da parte del Senato: sull'omissione di soccorso non si possono fare sconti. Questo è un tipo di reato, non saprei neanche se chiamarlo reato o in maniera più forte, ma certamente è un fatto bestiale, sul quale non ci può essere indulgenza. Può capitare la disgrazia, ma quando una persona, dopo una disgrazia, abbandona o omette il soccorso all'altra persona che è stata, come in questo caso, investita, si macchia di un reato che è veramente tra i più infami e tristi. Credo, quindi, sia necessario anche prevedere un provvedimento che renda giustizia a coloro che subiscono questi torti, non consentendo alcun beneficio a chi si macchia del reato di omissione di soccorso. È un segno di civiltà, signor Presidente, e lo dico anche al Governo: è un segno importante che dobbiamo dare, perché da questo punto di vista non esiste comunità civile che non sappia far rispettare le persone deboli che vengono, come in questo caso, travolte da disgraziati che niente hanno a che fare con le persone oneste che incontriamo tutti i giorni per strada. *(Applausi

per rivedere alcuni passaggi fondamentali che si sono svolti all'interno di quest'Aula. Intanto, esprimo solidarietà nei confronti del collega Esposito

giudizio - di giustificare l'atteggiamento di qualche squilibrato nel manifestare espressioni molto rudi, e conseguentemente non c'è giustificazione che possa tenere rispetto a coloro i quali si esprimono in modo non corretto e violento nei confronti non soltanto dei parlamentari ma di qualsiasi cittadino.

perché è vero quello che dice il senatore Zanda, ma non è vero che noi siamo liberi all'interno di questo Parlamento, e fuori da qui, di esercitare serenamente la nostra attività e di professare con grande forza le nostre idee, perché alcune *lobby*, e molte volte alcuni partiti, cercano di condizionare i parlamentari per portare avanti talune linee che molte volte sono in contrasto con l'interesse del Paese.

perché quando una persona all'interno di questo Parlamento, un senatore o un deputato, ha il coraggio di sostenere le proprie idee, ha il coraggio di schierarsi contro il partito nell'interesse del Paese, ci sono *lobby* e gruppi di giornalisti mediocri che operano al servizio di coloro i quali dettano le regole per delegittimare il Parlamento, e conseguentemente non dare la libertà al parlamentare di esprimere la propria idea! E chi vi parla è un parlamentare che è stato massacrato perché ha avuto il coraggio di esprimere liberamente il proprio modo di pensare! Allora, concludo, signor Presidente: mi fa piacere

Venerdì notte a Chiomonte è accaduto un fatto ripreso da tutte le televisioni nazionali, con immagini molto chiare. Da mezza Europa, come hanno testimoniato le presenze e i fermi della Polizia, si sono radunate circa 300 persone. Come mostrano le immagini, che penso vedano anche i colleghi del Movimento 5 Stelle, nette e chiare, questi 300 personaggi (io li ho chiamati delinquenti, e lo ribadisco) si sono organizzati con maschere antigas e con tutte le armi contundenti ed esplosive di cui dispongono (per fortuna non hanno ancora le bombe a mano) ed hanno annunciato e poi messo in atto un attacco, solo l'ennesimo, al cantiere TAV. Sapete cosa è successo questa volta, a differenza delle altre? Che la Polizia, invece di stare dentro il recinto e prendersi addosso bombe carta e razzi lanciati con dei mortai artigianali, ha deciso di svolgere la propria funzione ed è uscita in campo aperto. Vi indignate tanto per le manganellate, ma se domani mattina pensate di prendere a schiaffi un poliziotto in mezzo alla strada, cosa pensate che vi faccia? Che vi baci e vi abbracci? Se 300 teppisti che voi, purtroppo, legittimate con interventi come quelli che avete fatto in quest'Aula attaccano un cantiere, sono la legalità o la non legalità? Per me, la legalità sono quei ragazzi in divisa: poliziotti, carabinieri e finanzieri, che difendono lo Stato e usano gli strumenti che lo Stato ha messo a disposizione, che sono anche i manganelli. O pensate che dovrebbero usare le pistole? Io non lo penso: lacrimogeni e manganello. Gruppo M5S).* Dieci arrestati, di cui sette convalidati e tre no, tutti di Regioni diverse dal Piemonte, vi voglio segnalare, a dimostrazione che c'era il ritrovo dei centri sociali di tutta Italia, alla presenza in cantiere di due magistrati della procura della Repubblica di Torino, diretta da Giancarlo Caselli. Sono stati mandati lì preventivamente, perché era stato annunciato sui giornali pubblicamente, con l'intervista su «La Stampa», che ci sarebbe stato un attacco al cantiere, e hanno potuto vedere con i loro occhi quello che è successo. Allora faccio una domanda: la signora Marta da Pisa, che indossa una maschera antigas e va contro i poliziotti, si aspetta che i poliziotti la abbraccino?

Viene fermata come gli altri sette e viene portata al cantiere. Perché non ha immediatamente denunciato davanti ai magistrati di essere stata molestata? Perché non lo ha fatto? Per quale ragione ha atteso ventiquattrore e ha tenuto una conferenza stampa che è pubblica ed è su «Youtube», nella quale definisce la Polizia italiana «dei delinquenti»? Io ritengo che abbia usato il suo corpo per inventarsi una storia, perché non sapeva come giustificare la sua presenza al cantiere contro la Polizia.

Grazie,